*(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, questa interpellanza fu presentata all'indomani della presentazione del provvedimento sulle cosiddette liberalizzazioni, volute dal Governo, poi confluito in un provvedimento più ampio che,

agli atti parlamentari con il nome prima di Bersani-Visco e poi, vista la preminenza della parte fiscale su quella dedicata alle liberalizzazioni, con il nome Visco-Bersani. In quei giorni, leggemmo sui giornali che il

provenivano dall'Autorità garante, quella che per brevità viene designata come *Antitrust*. Leggemmo anche alcune dichiarazioni ed interviste del presidente di quell'autorità, il dottor Catricalà, che si compiaceva per l'intervento governativo. Ci vennero due preoccupazioni, entrambe espresse attraverso questa interpellanza. La prima fu una preoccupazione di ordine istituzionale. Il rapporto tra le Autorità indipendenti e il Parlamento è preminente rispetto a quello che può esistere tra

oltremodo grave, non foss'altro che per una questione di stile. È evidente che il Governo può prendere in considerazione le segnalazioni che l'Autorità *antitrust* fa al Parlamento; esse sono pubbliche e quindi anche a disposizione del Governo. Ci sembrava però di scorgere un rapporto particolare. Devo dare atto al presidente Catricalà di aver tenuto conto di questa preoccupazione, di aver risposto ad

della quale dovremmo farci carico tutti, Parlamento e Governo, ed è quella che concerne le modalità di raccordo e di comunicazione che devono esistere tra le Autorità indipendenti e il Parlamento. a me sembra insufficiente che questi modi di comunicazione si esauriscano in una sorta di manifestazione annuale

le liberalizzazioni servono ad aprire i mercati, a favorirne l'allargamento e, di conseguenza, a consentire a nuovi *players*, a nuovi attori

sviluppare un'opera di liberalizzazione. La ragione è semplice: è lì che si concentrano i grandi interessi economici ed è lì che, dunque, un'opera di liberalizzazione può creare

energia e gas naturali, trasporto ferroviario, secondo ciclo del sistema educativo d'istruzione, previdenza complementare (peraltro, oggi messa a serio rischio per un'avventuriera operazione sul TFR annunciata attraverso la finanziaria), affidamento dei lavori nelle concessioni pubbliche, servizi ambientali e gestione dei rifiuti; ma si potrebbe andare anche oltre, ricordando il trasporto urbano ed altri settori.

all'idea di società di cui l'attuale maggioranza è portatrice. Se così fosse, si cadrebbe in una contraddizione grave: non solo perché quel provvedimento verrebbe a mancare di equità,

signor Presidente, dal momento della presentazione dell'interpellanza ad oggi ci ha confermato in questi dubbi e in questi sospetti. sospetti. Altre liberalizzazioni sono state annunziate, ma, guarda caso, sempre negli stessi settori; altri comparti, dove interessi corporativi e blocchi monopolistici hanno conseguenze molto più serie sullo sviluppo economico del Paese, continuano invece ad essere ignorati, nonostante l'attività di segnalazione dell'*Antitrust* vada invece avanti.

Si citano, tra gli altri, i dati del *Fraser Institute*, che fa registrare questo *deficit* di competitività del nostro Paese. Sono naturalmente graduatorie fatte a livello internazionale, che possono anche essere discutibili per i parametri che vengono scelti, ma che certamente sono significative soprattutto nell'indicare un *trend* che dobbiamo tener presente. Ebbene, se è vero che l'Italia si trova oggi al 42° posto di tale graduatoria, devo tuttavia ricordare che purtroppo è proprio nel periodo tra il 2000 e il 2006 che si è registrato un forte peggioramento.

Anche la classifica del *World economic forum* ha un andamento simile, con un forte peggioramento nella graduatoria proprio negli ultimi cinque anni, dopo che nel quinquennio precedente si era faticosamente risaliti. Potremmo dire

Del resto, senatore Quagliariello, lo dico non per spirito polemico, ma per oggettiva constatazione, se lei giustamente può ricordare un così lungo elenco di segnalazioni dell'*Authority*

impegno preciso. Non sono state condotte politiche di liberalizzazione in settori strategici, semmai, come è avvenuto nel campo dell'energia, sono state ritardate liberalizzazioni che il Governo precedente aveva avviato. Comunque, preferisco cogliere l'aspetto positivo dell'interpellanza, perché, in via generale, condividiamo l'importanza strategica per la competitività del nostro Paese di riuscire a mettere in campo azioni coerenti di liberalizzazione. Potrei rinviare al DPEF, a questo documento fondamentale della programmazione, che da pagina 92 a pagina 96, individua proprio le motivazioni politiche ed economiche, i settori, i metodi e le priorità di intervento per promuovere la concorrenza e migliorare la condizione dei consumatori. Devo contestare che il decreto-legge n. 223 del 2006 abbia avuto una volontà La lettura dell'insieme dei settori toccati da quel provvedimento consente, infatti, di vederne la rilevanza strategica per l'incidenza nell'intero campo dei servizi. Con quest'ottica vanno valutate le misure, che incidono anche sulla vita quotidiana dei cittadini, riferite alle libere professioni, alla distribuzione commerciale, ai farmaci, alla panificazione, ai taxi, ai notai, alle assicurazioni auto, ai prezzi dei prodotti agroalimentari, ai conti correnti bancari, ai poteri dell'Autorità di vigilanza che vengono rafforzati, appunto, non certo perché la interpretiamo - e lungi da noi avere questa idea così rozza una sorta di ufficio studi del Ministero. Quindi, non si è trattato di un intervento selettivo, ma generale. Con il decreto-legge ora citato sono state eliminate ben quattordici restrizioni alla concorrenza, che hanno recepito altrettante puntuali segnalazioni che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come lei, senatore Quagliariello, giustamente richiama, aveva ripetutamente formulato nel corso delle precedenti legislature; alcune specifiche norme del decreto‑legge hanno altresì consentito all'Italia di superare favorevolmente quattro procedure d'infrazione comunitaria che ormai erano giunte davanti alla Corte di giustizia. Naturalmente, siamo ben coscienti che questo primo provvedimento affronta solo una parte dei problemi del Paese in questo settore e abbiamo confermato la volontà di proseguire in un'azione politica incisiva di liberalizzazione non solo a parole, non solo con impegni politici, ma anche con atti legislativi concreti. Sono infatti all'attenzione del Parlamento un disegno di legge sui servizi pubblici locali, un disegno di legge contenente una delega per la liberalizzazione nel settore energetico, un disegno di legge sull'azione collettiva di tutela del consumatore e le norme attuative delle nuove disposizioni per la tutela del risparmio. Dunque, pensiamo che vi siano occasioni importanti per poter misurare la capacità riformista del Governo e la capacità del Parlamento, direi nel suo insieme, di raccogliere questi stimoli. Finora abbiamo visto autorevoli esponenti dell'opposizione porsi alla guida delle proteste di quei settori che hanno cercato di opporsi alle necessarie novità legislative: ci avete chiesto di essere meno liberalizzatori, non più liberalizzatori. Mi auguro che d'ora in poi, anche sulla scorta delle sollecitazioni che sono contenute nell'interpellanza, possiamo ricevere anche dall'opposizione stimoli per fare di più e non di meno, in questo campo. Pensiamo che serva al futuro del Paese: serve alle giovani generazioni che hanno il diritto di avere le stesse opportunità di affermazione che hanno avuto le generazioni precedenti.

fortemente discriminatorie nei confronti di una parte della popolazione, di una parte dei cittadini; vi chiediamo inoltre di non favorire solamente quegli attori sociali che sono più vicini alla vostra visione ideologica e dei vostri interessi

discutere di cosa significhi tutela della concorrenza: se continuare a privilegiare un'ottica orientata al mercato, *market oriented*, come dice la letteratura anglosassone, oppure indirizzarsi a politiche di tutela e di concorrenza indirizzate verso il consumatore. è una differenza fondamentale tra questi due approcci e ho l'impressione che il Governo di centro-sinistra stia sempre più privilegiando il primo dei due. Si comprendono così anche alcuni interventi impropri e a gamba tesa compiuti da questo Governo o dai collaboratori di questo Governo in ambiti nei quali invece si sarebbe dovuto lasciare assoluta libertà al mercato. Se quegli interventi fossero venuti da un Governo di centro-destra avreste fatto la rivoluzione, e giustamente. Così si possono comprendere anche le finte liberalizzazioni che state cercando di fare - vedo che nel banco del Governo c'è anche il sottosegretario Vimercati nell'ambito della televisione, spacciando per legge di liberalizzazione una legge punitiva, che premia i monopoli su alcune piattaforme solamente perché vi sono attori più vicini al Governo e punisce invece fortemente altri attori che sono più vicini al consumatore, creando un danno

Ho l'impressione che gli spazi per una politica riformista in senso liberale e di liberalizzazione, purtroppo, per questo Governo si sono ristretti.

precedenza che avete ritenuto di accordare, sempre e in ogni caso, al sindacato. Avete fatto una finanziaria nella quale sono stati toccati gli poveri e ricchi - mi consenta questa semplificazione polemica - ma, d'altra parte, è stato concesso al sindacato tutto ciò che voleva. Basta guardare il capitolo della pubblica amministrazione

in questi ultimi giorni, non saranno altro che le prime di una lunga serie, se il Governo continuerà a operare in questo senso.

Per quanto riguarda, invece, la mia interpellanza, attendo la risposta che fornirà il Governo per poi intervenire nel merito.

è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2003, il presidente della Società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN) è stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari. Con successivi provvedimenti lo stato di emergenza inerente alla suddetta attività è stato, poi, prorogato fino al 31 dicembre 2006. Il mandato del commissario delegato - come giustamente è stato anche richiamato nell'interpellanza - era circoscritto alla messa in sicurezza dei materiali nucleari e alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari, nonché degli impianti del ciclo del combustibile nucleare e dei depositi di materie radioattive dislocati nei territori delle Regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte. In particolare, la suddetta ordinanza del 2003 ha previsto, all'articolo 2, un elenco di norme che potevano essere derogate. In questo contesto, il commissario delegato, dal 2003 ad oggi, ha effettuato una serie di interventi di messa in sicurezza fisica degli impianti e delle infrastrutture contenenti materiali nucleari nei vari siti nazionali; ha inoltre predisposto i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, riferendo sullo stato di avanzamento dei lavori sia alla commissione tecnico-scientifica, sia al Dipartimento della protezione civile. Lo stesso commissario delegato ha, tuttavia, avviato anche alcune iniziative che, per loro natura, comportano tempi molto lunghi di realizzazione, che vanno oltre quelli tipici di un provvedimento di emergenza. Rientrano tra questi ultimi interventi quelli che il commissario delegato definisce «criticità residue» in una relazione fatta alla commissione tecnico-scientifica.: Gli organi competenti alla verifica ambientale e gli enti locali coinvolti hanno fatto, quindi, rilevare che le predette attività avrebbero dovuto essere gestite, sia in fase autorizzativa che in fase di realizzazione, non in «emergenza», ma seguendo le normali procedure previste dalle vigenti leggi. In conclusione, il commissario delegato ha senz'altro contribuito a risolvere i problemi di sicurezza; d'altra parte, approssimandosi il termine di scadenza fissato al 31 dicembre 2006 e in considerazione dell'avvenuta definizione e attivazione delle misure di sicurezza, il Governo intende riconsiderare la situazione, alla luce della necessità di recuperare le ordinarie competenze e procedure di gestione e di riallacciare chiari e trasparenti rapporti di leale collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti e con gli enti locali coinvolti, al fine di favorire sia un più adeguato livello di efficienza degli interventi ancora da effettuare, sia di favorire la trasparenza delle operazioni e la piena informazione delle popolazioni interessate.

La raccomandazione è quella di cambiare l'amministratore delegato. Tale raccomandazione è molto sentita e motivata dal fatto che, se questo orientamento del Governo fosse stato pronunciato e maturato nel momento dell'interpellanza, probabilmente avremmo evitato altri elementi negativi. Segnalo due elementi negativi. Rispetto alla messa in sicurezza e alla cura degli impianti, temo che si sia più seguita la linea degli investimenti e delle speculazioni finanziarie, nelle quali abbiamo lasciato 3 milioni di euro di disavanzo, una non cura della famosa messa in sicurezza, tanto che sia l'impianto della Casaccia, sia l'impianto Eurex di Saluggia hanno manifestato delle fughe,

L'altro elemento negativo riguarda il materiale radioattivo. Si tratta di materiale che va in Francia e viene lavorato in Francia; non facciamo quindi che rinunciare ad un problema che abbiamo. È comprensibile, infatti, che collocare sul territorio materiale radioattivo, per quanto in sicurezza e con impianti moderni, possa incontrare

Signor Presidente, in via generale, si osserva che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevedeva, all'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, che l'Enel spa costituisse una società separata per lo «smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti». In data 31 maggio 1999 l'Enel spa ha costituito la SOGIN spa, il cui statuto, all'articolo 4 («Oggetto della società»), afferma che la società ha per oggetto l'esercizio delle attività relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e le attività annesse e conseguenti. La società, inoltre, può operare sia in Italia che all'estero e svolgere qualsiasi attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il perseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo, il recupero e la valorizzazione dei siti in cui sorgono le centrali elettronucleari e l'adeguamento di sicurezza delle centrali medesime. La società può, inoltre, svolgere attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizi in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale. A questo ultimo riguardo, l'articolo 1, comma 103, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ha imposto alla società SOGIN di svolgere le attività di prestazione di servizi per conto terzi in regime di separazione contabile. Con la legge 31 luglio 2005, n. 160, è stato, poi, ratificato l'accordo di cooperazione tra Italia e Federazione Russa per lo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dal servizio e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato. L'accordo di cooperazione individua nella SOGIN il soggetto attuatore di parte italiana, facendo seguito ad intese definite nel corso del vertice del G8 di Kananaskis del giugno 2003. L'accordo di cooperazione, che riguarda l'arco temporale di un decennio, prevede un impegno finanziario italiano di 360 milioni di euro e quindi il conferimento di risorse alla società SOGIN spa, ma solo per le attività successive al mese di agosto 2005. È chiaro, peraltro, che le attività di prestazione di servizi per conto terzi svolte dalla società SOGIN S.p.A. non possono avvalersi delle risorse finanziarie messe a disposizione della stessa società come componente della tariffa elettrica, per la gestione dei materiali nucleari e lo smantellamento degli impianti del programma nucleare italiano. In tale quadro, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 25 maggio 2006, n. 106 non ha riconosciuto alla SOGIN S.p.A. l'aumento, rispetto al valore medio annuo del triennio precedente, degli oneri nucleari per le attività svolte nel 2005, relativi sia alla voce *«project management»* degli impianti (1,7 milioni di euro), sia alla voce coordinamento e servizi generali (1,3 milioni di euro), per un totale di 3 milioni di euro: ai costi delle attività di servizio non riconosciuti attraverso le tariffe elettriche la società ha dovuto far fronte con il fondo di dotazione. In ogni caso, nella sua posizione di organo con compiti di indirizzo, il Ministero dello sviluppo economico intende intervenire affinché la società SOGIN S.p.A. svolga in modo regolare, tempestivo ed efficace il suo mandato, con particolare riferimento alla missione assegnata dalla legge. È quindi intenzione del Ministero verificare la correttezza delle regole e delle procedure adottate nella gestione della società, con particolare riferimento alle spese e imputazioni di costi che non appaiano fondate. Il Governo sta, inoltre, valutando le possibili iniziative di riordino dei profili funzionali e istituzionali e di assetto gestionale e organizzativo della società. considerazioni precedentemente fatte. Nel merito: proprio la vicenda dei sommergibili nucleari russi, affrontata dalla trasmissione *Report*,

È proprio in quella vicenda che abbiamo perso la faccia, perché i sommergibili sono ancora là, e rimesso dei soldi per le operazioni fatte dalla SOGIN

se ci fosse stato un occhio più attento, al tempo dell'interpellanza, si sarebbe probabilmente colto l'elemento importante, ovvero che un'operazione di questo tipo, di valenza internazionale, vedeva l'Italia coinvolta,

dice san Tommaso d'Aquino, che era un genio del senso comune, che chi vuole il fine deve volere anche i mezzi che conducono al fine. Il Governo Prodi, invece, vuole la ferrovia Lione-Torino, lo ha dichiarato in ogni modo, con grande convinzione - lo ha detto il ministro Di Pietro, lo ha detto il presidente del Consiglio Prodi, lo hanno detto tutti - e io ci credo perché, come diceva Shakespeare, Prodi è uomo d'onore. fulminante. BUTTIGLIONE *(UDC)*. Ci credo davvero, e lei ammetterà che personaggi di tale rilievo meritino qualche riferimento letterario. Tuttavia, mi sembra che non si vogliano i mezzi che consentono di realizzare il fine, ovvero di costruire la ferrovia ad alta velocità e ad alta capacità: c'è stata pure una polemica sul concetto di alta velocità e di alta capacità, ma dove c'è

perché l'Unione Europea giustamente si concentra sulle tratte transfrontaliere. Credo sia difficile che l'Italia possa finanziare per intero quest'opera rinunciando a tale contributo.

Questo contributo deve essere inserito nella pianificazione finanziaria 2007-2013 e a questo fine è necessario che l'Italia prenda le sue decisioni relative alla realizzazione dell'opera,

Nonostante il meritorio sforzo del ministro Di Pietro in occasione di un recente convegno per rassicurare in tal senso, non ci crede nessuno. Esistono anche alcune dichiarazioni semiufficiali che

per definire il percorso della ferrovia e le modalità di realizzazione dell'opera, ha scelto il metodo della Conferenza dei servizi, rinunciando a far uso della cosiddetta legge grandi opere, che consente una procedura semplificata

certamente dialogo, ma il dialogo deve condurre alla decisione e l'uomo di Stato è il decisore, colui che alla fine del dialogo si prende la responsabilità della decisione

la scelta di questo metodo di decisione assegna a ciascuno dei Comuni che partecipano alla Conferenza stessa un diritto di veto. Anche se c'è chi ammette in sede teorica, dal punto di vista giuridico, come ha fatto una volta meritoriamente il ministro Bersani, che il Ministro si può prendere la responsabilità di decidere,

Quindi, ognuna delle componenti, ognuno dei Comuni, ma anche ognuna delle forze della maggioranza ha un diritto di veto. É inoltre ben noto che alcuni Comuni ed alcune componenti della maggioranza hanno dichiarato a gran voce di essere intenzionati ad esercitare questo diritto di veto. Si capisce allora perché a Bruxelles nessuno creda che si arrivi a realizzare la ferrovia Lione-Torino. Non ci si dica che state utilizzando questo tempo per acquisire ulteriori informazioni

Da un tempo di poco inferiore si dialoga con le popolazioni e non esiste il tempo per studiare effettivamente percorsi alternativi, salvo varianti minimali che certamente non sono in grado di portare a far cambiare idea a coloro che sono oggi contrari. Peraltro, di percorsi alternativi si parla. Un giorno si dice che l'alta velocità passerà da Genova e il Presidente della Regione Liguria ha già dichiarato di essere pronto in tal senso. Il giorno seguente passerà più per Genova, ma per Val Sangone e il terzo giorno per la Svizzera e la Valle d'Aosta. In realtà, siccome non sono cose che si improvvisano ma che richiedono preparazione e studi di lungo periodo,

solo grazie all'impegno del Governo Berlusconi, del quale avevo l'onore di fare parte come Ministro delle politiche comunitarie - ho avuto qualche parte anche nelle trattative che hanno portato a tale decisione - è la Strasburgo-Stuttgard-Salzburg-Vienna. Questa alternativa, che passa sopra le Alpi, taglierebbe l'Italia fuori dal sistema delle reti TEN (*Trans-European Networks*), isolandoci dall'Europa e condannando il Paese al declino economico.

perché se Torino vuole mantenere la vocazione di città manifatturiera - e può e deve mantenerla - può farlo facendo affluire da tutto il mondo componenti ed elementi a cui dare il tocco finale con il lavoro altamente altamente qualificato dei torinesi e ridistribuendoli poi in tutto il mondo: un'efficiente rete logistica è la condizione indispensabile perché Torino mantenga una vocazione industriale e manifatturiera. Inoltre, noi avremmo o avremo - avremo o avremmo? Chi lo sa, temo di dover dire avremo - a breve scadenza una crisi dei valichi alpini. Infatti, il traffico su ruota, attraverso i valichi che conducono in Francia, è già intensissimo, insopportabile, pericoloso per la salute delle valli alpine; vorrei dirlo a chi è contrario alla Lione-Torino per ragioni ecologiche: il traffico autostradale sui valichi alpini è rovinoso. Lo dico qui, fra di noi, sperando che non mi sentano in Francia, perché a suo tempo lo dicevano i francesi per spiegarci il motivo per cui un giorno sì e l'altro pure chiudevano a turno uno dei valichi alpini per ridurre il danno. Il traffico ma è destinato ad aumentare in maniera esponenziale nei prossimi anni: possiamo calcolare nell'arco di un decennio il raddoppio o più del raddoppio degli attuali volumi di traffico. Proprio per questo la Francia aveva già cominciato a proteggersi, chiudendo l'uno o l'altro dei valichi. Noi portammo allora il problema davanti alla Commissione europea, sostenendo che non si trattava di un problema italo-francese, ma di un problema europeo, perché veniva negato agli operatori italiani il diritto di libera circolazione delle merci in Europa. Riuscimmo ad argomentare con efficacia questa posizione davanti ai commissari europei Bolkestein e Loyola de Palacio, due grandi Commissari, dotati anche di grande sensibilità verso l'Italia, severi, severi, ma giusti e disponibili a capire le nostre ragioni. Con il loro aiuto e con l'aiuto dell'allora presidente della Commissione europea Romano Prodi, riuscimmo a costringere, o a convincere, la Francia a riaprire i valichi. Tuttavia, dell'accordo raggiunto

La Lione-Torino triplica così i volumi di traffico delle merci trasportabili e, pur non consentendo in verità di diminuire di molto il traffico attuale, permette certo di assorbire gli aumenti prevedibili di traffico dei prossimi anni. Se viene meno la Lione-Torino, si riapre inevitabilmente il contenzioso dei valichi alpini e non vorrei essere nei panni del Ministro *pro-tempore* delle politiche comunitarie o dei trasporti e infrastrutture che dovrà andare a trattare con i francesi: ci chiuderanno i valichi. i valichi. In alternativa, o in contemporanea, avremo un danno irreparabile per l'ambiente alpino, contrario anche alla Convenzione delle Alpi che il Governo italiano ha sottoscritto. È nostra impressione che il Governo non voglia decidere per non rischiare spaccature all'interno della maggioranza. Rendo omaggio al sindaco di Torino Chiamparino che, invece, nel corso di un violento dibattito nel Consiglio comunale di Torino, alla fine ha preso il coraggio a due mani affermando che, dovendo scegliere tra

il tempo di decidere è adesso. Chiediamo al Governo impegni precisi e tempi certi per la loro realizzazione.

in via preliminare si deve confermare che la realizzazione della nuova tratta ferroviaria Torino-Lione riveste carattere prioritario. Ciò doverosamente premesso, si ricorda che, alla luce delle proteste delle popolazioni della Val di Susa, che avevano, di fatto, bloccato la prosecuzione delle attività esplorative relative al progetto, il Governo, appena insediatosi, ha tenuto una riunione lo scorso 29 giugno presso la Presidenza del Consiglio con la Regione Piemonte ed alla presenza degli enti territoriali. Ciò al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle comunità locali nel procedimento autorizzativo dell'opera. In tale riunione è stato deciso, pertanto, di stralciare tale procedimento autorizzativo dalla legge obiettivo e di ricondurlo alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 81 del decreto Il CIPE ha successivamente confermato tale decisione in sede di approvazione dell'allegato infrastrutture al DPEF relativo al periodo 2007-2011. Per quanto attiene alle osservazioni avanzate dai senatori interroganti, si riferisce che il coordinatore europeo per il progetto prioritario n. 6 (Lione-Torino‑Milano-Trieste-Lubiana-Budapest), nella propria relazione annuale di attività ha illustrato le proposte indicative di sostegno comunitario che lo stesso coordinatore intende presentare alla Commissione europea nell'ambito della programmazione finanziaria 2007-2013. Lo stesso coordinatore ha, in proposito, ritenuto che la priorità del cofinanziamento comunitario, a titolo del bilancio 2007-2013, dovrebbe andare alla realizzazione delle sezioni transfrontaliere, secondo la ripartizione di seguito riportata: un sostegno equivalente al 20 per cento del costo della sezione transfrontaliera franco-italiana pari, per il periodo 2007-2013, a circa 1 miliardo di euro (condizione di tale finanziamento è la garanzia, da parte delle autorità italiane, di fare il possibile, nei tempi più rapidi, per trovare soluzioni alle difficoltà incontrate nella Val di Susa); un sostegno pari al 10 per cento del costo totale delle sezioni di accesso francesi e italiane alle gallerie di base, pari a circa 237 milioni di euro per la parte italiana; un sostegno fino al 50 per cento per la prosecuzione degli studi della sezione italo-slovena e delle sezioni tra Divaca e Budapest. Relativamente ai quesiti posti dai senatori interroganti in merito alla posizione del Governo rispetto alle valutazioni contenute nella relazione annuale del coordinatore europeo e alle iniziative che si intendono assumere per consentire l'utilizzazione dei fondi comunitari, si conferma che sono in corso le occorrenti valutazioni ed analisi con l'obiettivo di definire in tempi rapidi, congiuntamente alla parte francese, una proposta comune per la richiesta del finanziamento dell'opera. per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dallo stesso coordinatore in merito all'opposizione al progetto di una parte della popolazione della Val di Susa ed alle conseguenti ripercussioni sul calendario di realizzazione, si conferma che, proprio allo scopo di corrispondere all'impegno richiesto relativamente ai tempi di conclusione delle procedure appropriative, è già in corso di affidamento lo studio di impatto ambientale dell'intera opera da parte di LFT, che è promotore dell'opera. Come precisato nella precedente lettera, il SIA costituisce l'elaborato di riferimento, attraverso anche l'esame di vari e differenti scenari realizzativi delle analisi costi-benefìci, ai fini della valutazione di impatto ambientale. Una volta conclusa la valutazione di impatto ambientale, la conferenza di servizi ex articolo 81 del suddetto decreto potrà pronunciarsi in via definitiva. Giova precisare, in ogni caso, che a seguito dei disordini verifìcatisi nella Val di Susa, sono state avviate indagini giudiziarie, tra l'altro, per danneggiamenti prodotti alle attrezzature di cantiere. Tali indagini hanno portato al sequestro dell'area oggetto degli eventi e delle stesse attrezzature che, su disposizione della magistratura, sono state trasportate in depositi giudiziari. Proseguono, inoltre, i lavori della Conferenza dei servizi, nuovamente riunitasi il 12 ottobre ultimo scorso ed alla quale hanno preso parte, tra l'altro, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i rappresentanti della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia e della Comunità Montana Alta Valle Susa, nonché i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati. In quella sede, le Amministrazioni e gli enti intervenuti hanno esposto le proprie osservazioni sugli elaborati progettuali trasmessi da L.T.F. ed R.F.I. in ottemperanza a quanto deciso dalla Conferenza nella riunione del primo agosto ultimo scorso. In particolare, la Regione Piemonte, a mezzo dei propri rappresentanti, con osservazioni condivise dalla Provincia di Torino, ha fatto presente di ritenere che lo sviluppo complessivo del tracciato soddisfi le condizioni generali, pur ravvisando la necessità di alcuni approfondimenti per quanto attiene al progetto della tratta internazionale. Il Presidente della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia ha, invece, richiesto, a nome di trentasette consigli comunali che hanno manifestato parere contrario sugli elaborati progettuali delle due tratte, quella nazionale e quella comune italo-francese, la sospensione della Conferenza dei servizi e la convocazione del Tavolo politico per individuare le modalità operative e di funzionamento dell'Osservatorio tecnico. Tale richiesta, cui ha aderito anche il Presidente della Comunità Montana Alta Valle di Susa, non è stata ritenuta accoglibile dal Ministero delle infrastrutture che ha sottolineato, da un lato, la natura istituzionale ed amministrativa della Conferenza dei servizi, quale istituto regolamentato da specifiche normative che ne disciplinano tempi e modalità e, dall'altro, la sua rilevanza autonoma rispetto ad altre sedi (Osservatorio tecnico/Tavolo politico), aventi natura e finalità diverse. Si è, inoltre, ribadito, nei confronti degli enti locali che hanno preso parte alla riunione, l'assoluta rilevanza dell'opera quale occasione di sviluppo economico e sociale dei territori interessati, fornendo, in ogni caso, assicurazioni sull'inesistenza di preclusioni in merito alla possibilità di esaminare diverse ipotesi progettuali. Preme sottolineare, poi, che il Commissario straordinario del Governo per «il coordinamento di tutti gli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico relativi all'asse ferroviario Torino-Lione» architetto Mario Virano, intervenuto alla riunione, ha rimarcato l'utilità dello strumento della Conferenza dei servizi e del relativo metodo procedimentale, esprimendo la propria condivisione in ordine allo stralcio dell'opera dalle procedure approvative previste dalla legge obiettivo ed alla sua sottoposizione a quelle ordinarie. Si fa presente, infine, che è stata fissata per il giorno 9 novembre prossimo venturo, la riunione del cosiddetto Tavolo politico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la prossima riunione della Conferenza dei servizi è stata programmata per il giorno 13 novembre prossimo Per quanto riguarda, infine i tempi previsti per il completamento dell'*iter* approvativo del progetto si prevede l'ultimazione dello Studio di impatto ambientale -SIA - entro l'aprile del 2007, la conclusione della procedura di

si potrebbe giungere all'ipotesi di diverse soluzioni progettuali, che prenderebbero altro tempo e che farebbero annullare conseguentemente l'opera. Procedendo in questo modo, riteniamo che le cose non siano chiare, come ben ha detto all'inizio il senatore Buttiglione:

tutto viene dilatato e prolungato. Alla fine, si andrà troppo per le lunghe e non si arriverà alla conclusione probabilmente di niente! di niente! Questo sarà un ulteriore danno, il danno vero per la città di Torino, per il Piemonte, per l'intero sistema economico di trasporto del Nord d'Italia. Questo Governo se ne assume la responsabilità;

si continua ad essere ostaggi di quelle frange estreme, di quell'ambientalismo estremo che non può che portare alla *impasse* sia delle grandi opere che dell'intera nostra comunità ed economia.

di informazioni che, per la verità, erano già a nostra conoscenza e che non costituivano il tema dell'interrogazione. Sappiamo anche noi quel che succede a Bruxelles. Senza offesa, mi veniva in mente il mio grande maestro Augusto Del Noce, che usava dire che la filosofia analitica dimostra in modo sempre più rigoroso proposizioni sempre più irrilevanti. Lei ci ha dimostrato in modo rigoroso proposizioni che non attengono al nostro problema. Diceva anche Del Noce che l'oscurità dell'espressione non sempre, ma molte volte è sintomo dell'incertezza del pensiero. Ora, lei è persona garbata, competente, intelligente ma non ha dietro il supporto politico necessario per parlare con chiarezza. Quel che noi volevamo sapere è: il Governo ritiene che, in sede di Conferenza di servizi, alla fine ha il diritto di prendere una decisione, anche qualora permanesse il veto di 37, 38, 39 o 40 Comuni che siedono in quella consesso, o accetta o accetta l'interpretazione secondo la quale, in mancanza dell'accordo, tutto si deve fermare? Questo non è chiaro. Non è sufficiente dire che non bisognava aprire il tavolo politico, perchè i tavoli politici sono sempre aperti: ogni giorno ci incontriamo, ci telefoniamo, ci parliamo. Il Governo intende agire o no? Mi consenta anche di dire che credo che alcune cose da lei dette non siano del tutto esatte. Lei ha parlato del fatto che, in sede europea, sono pronti ad inserire la TAV Lione-Torino nel piano finanziario 2007-2013, in cambio della garanzia che il Governo farà il possibile nei tempi più rapidi! No; non vogliono la garanzia che il Governo farà il possibile, vogliono la garanzia che il Governo farà; non farà il possibile per fare, ma farà. Le pare possibile che si inserisca nella programmazione finanziaria senza una certezza, che derivi dal compimento di atti e che ci si fidi una promessa? Lei non lo crede: conosce troppo bene le procedure europee per immaginare che questo possa essere vero; però, l'ha detto. E poi, è in corso lo studio dell'impatto ambientale: qui, per la verità, i partecipanti alla Conferenza dei servizi qualche ragione ce l'hanno,

consentitemi ancora di rivolgere un memore pensiero all'imperatore Napoleone, non in quanto grande generale - perché questo è un aspetto della sua attività che suscita, giustamente, perplessità di carattere morale grande fondatore del diritto amministrativo. Ci ha insegnato, infatti, che esistono i diritti e gli interessi legittimi e che quando c'è un bene comune da realizzare, davanti ad esso non esistono diritti, ma solo interessi legittimi che danno luogo al diritto al risarcimento, ma non a quello di impedire l'opera. Il Governo condivide questa idea? È disposto ad agire sulla base di questa antica e consolidata tradizione del diritto amministrativo, per altro disattesa da non poche recenti sentenze dei nostri TAR?

Di nuovo: ma sappiamo cosa vuol dire realizzare un'alternativa di percorso che non sia lo spostamento di qualche centinaia di metri? Ma pensiamo davvero che in quel contesto orografico vi siano le condizioni per significative alternative di percorso? Siete consapevoli del fatto che state tentando semplicemente di guadagnare tempo, ma, alla fine, questo finisce? E se il tempo finisce senza una decisione, forse avrete salvato l'unità della vostra coalizione posto che questa non salti in aria su altri scogli, per altri motivi, prima di arrivare a quel momento - ma l'opera non si farà, e sarà un danno irrimediabile per la città di Torino, per il Piemonte e per tutta l'Italia.

Signor Presidente, innanzi tutto, per quanto attiene alla legittimità della nomina del dottor Risoli a componente del Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC), l'articolo 13, comma 12, del vigente Statuto della Fondazione

Tale disposizione prevede una valutazione di merito da parte del Consiglio generale in ordine ai requisiti dei candidati alla suddetta carica, in linea con il pieno riconoscimento dell'autonomia delle Fondazioni operata dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e dalla Corte costituzionale, con le sentenze nn. 300 e 301 del 2003. L'Autorità di vigilanza, quindi, non potrebbe sovrapporre la propria valutazione a quelle di merito espressamente rimesse all'autonomia del Consiglio, salvo il caso di palese irragionevolezza o di motivazione carente delle medesime. Sulla base degli elementi presentati, il caso del dottor Risoli non sembra rientrare in quest'ultima fattispecie, non potendosi ritenere astrattamente irragionevole l'interpretazione che il requisito di «esperto nel settore sanitario» non si riferisca alle sole persone che esercitano la professione sanitaria. Per quanto concerne la legittimità della nomina a componente del Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo del signor Falco, si premette che la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 301 del 2003, pur riconoscendo come «storicamente indiscutibile» il collegamento delle Fondazioni bancarie «con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine», riconosce in capo agli enti territoriali esclusivamente «un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo», potere che si esaurisce con il suo esercizio e non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati, al fine di superare il «rischio ... di trasformare le Fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali». Inquadrato il potere di nomina in capo all'ente territoriale, occorre verificare se lo stesso sia stato correttamente esercitato dal Comune di Borgo San Dalmazzo. A tal fine, è necessario interpretare il disposto dell'articolo 13 dello Statuto della Fondazione nella parte in cui prevede che il candidato proposto alla nomina dal suddetto ente locale sia scelto «tra cittadini residenti, da almeno tre anni, in un Comune della zona di Cuneo». Tale disposizione - nella sua formulazione letterale - non sembra presentare elementi idonei ad escludere che la dizione «zona di Cuneo» non comprenda anche il Comune che connota la zona medesima. Un'uguale espressione è, del resto, utilizzata nella lettera a) del medesimo articolo, in relazione al potere di nomina dell'amministrazione comunale di Cuneo. Pertanto, appare corretto ritenere - anche alla luce delle disposizioni del citato statuto della fondazione - che il citato ente territoriale abbia correttamente individuato nella persona designata quella più idonea a rappresentare la realtà territoriale, nella quale la propria comunità è inserita. In merito, infine, al presunto profilo di illegittimità delle nomine dei signori Falco e Oddero, fondato sulla considerazione che si tratterebbe dello svolgimento del terzo mandato consecutivo, il disposto dell'articolo 13, comma 6, del citato statuto, prevede che: «I componenti il Consiglio Generale durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo». Tale disposizione - si afferma nell'interrogazione in esame - dovrebbe prevalere sul disposto dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 150 del 18 maggio 2004, in quanto quest'ultimo prevederebbe una mera facoltà per le fondazioni di computare o meno il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del suddetto regolamento: la volontà dell'«estensore dello Statuto ... doveva essere esplicata con una disposizione specifica», la cui mancanza testimonierebbe la volontà di non avvalersi della suddetta facoltà; tale interpretazione da parte dell'interrogante non però appare condivisibile alla luce della *ratio* posta alla base della disposizione regolamentare in esame. Riprendendo quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere consultivo sullo schema del suddetto decreto ministeriale n. 2680 del 2004, deve ritenersi che tale norma, infatti, «appare giustificata dalla estrema incertezza del regime che ha caratterizzato il periodo in questione, nonché dalla limitazione» - ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale - «dell'attività di questi organismi ai soli atti di ordinaria amministrazione». Bisogna, poi, ricordare che, in riferimento all'autonomia riconosciuta alle fondazioni dalla legge (articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999) e dalla Corte costituzionale con le sentenze, già richiamate, nn. 300 e 301 del 2003, alla luce delle disposizioni costituzionali in materia di «formazioni sociali», non è precluso al legislatore di conformare la medesima autonomia nel caso in cui vi sia la necessità di tutelare esigenze inderogabili, come quelle richiamate. Il comma 4, dell'articolo 7, del decreto ministeriale n. 150 del 18 maggio 2004, deve essere quindi interpretato come applicabile a tutte indistintamente le fondazioni, senza necessità di una disposizione statutaria di recepimento. Peraltro, la fondazione, alla luce del principio di autonomia garantito in generale alle fondazioni e delle valutazioni circa l'interesse della fondazione, in relazione alla propria operatività istituzionale, avrebbe potuto decidere di non avvalersi del suddetto comma 4. Risulta, però, imprescindibile che tale scelta da parte della fondazione fosse compiuta in modo espresso, mediante un'apposita norma statutaria transitoria approvata dai propri organi, al fine di attuare l'inderogabile tutela degli interessi dei terzi, che vedrebbero altrimenti posta nel nulla una propria legittima aspettativa, se non un proprio diritto, nonché per motivi di trasparenza nei confronti dei soggetti statutariamente chiamati a designare i componenti degli organi. Per quanto riguarda, invece, il diritto di accesso all'atto di nomina, a cui è stato opposto dagli organi della fondazione un diniego verbale, deve richiamarsi l'attenzione sulla corretta qualificazione della natura giuridica delle fondazioni bancarie, sancita dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, secondo il quale le stesse «sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti». Pur essendo, quindi, «continuazione di enti pubblici», il riconoscimento legislativo della natura privata delle medesime - avallato anche dalle più volte richiamate sentenze della Corte costituzionale - preclude la soggezione delle medesime alla normativa in materia di accesso. Alla luce delle suddette motivazioni, non sembrano sussistere elementi che possano indicare che siano state compiute delle irregolarità nella procedura di nomina del consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, essendo stata data corretta attuazione alle disposizioni statutarie che regolano il procedimento di nomina del suddetto organo.

delle motivazioni che egli ha addotto - peraltro richiamando una serie di considerazioni che avevo svolto nell'interrogazione

si sia limitata nel primo caso, cioè quello della nomina del dottor Risoli, a interpretare in modo corretto la sussistenza dei requisiti, così come del ha fatto l'organo statutario che ha recepito le nomine. Come ho peraltro scritto nell'interrogazione, se è vero che non è necessariamente un esperto in materia sanitaria un medico o comunque chi si interessa direttamente di tale attività, diventa difficile - e facevo un esempio in che un medico sia esperto in ingegneria. Prendo comunque atto che il Ministero ha rinunciato alla sua facoltà di controllo. Per quanto riguarda, invece, la vicenda del dottor Falco, credo di aver argomentato le ragioni per le quali le quali è stata in questo caso perpetuata la nomina. Avendo egli lucrato già la nomina attraverso la designazione prima del Comune di Cuneo ed essendo stato per ben due mandati già nel Consiglio generale della Fondazione, della Fondazione, l'*escamotage* è stato quello di farsi designare da un Comune limitrofo, tenendo conto che il meccanismo, come è stato spiegato, è a rotazione.

maggiore nei confronti della generalità dei cittadini, perché se è vero che sono delle fondazioni di diritto privato, come è stato ricordato, la

di una fondazione bancaria che ha un patrimonio di circa 4.000 miliardi di vecchie lire e che esercita la sua attività nell'interesse dei cittadini.

In relazione all'atto parlamentare in esame, si ritiene opportuno ricordare che non rientra tra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti. Tali aspetti rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione e del direttore generale della società ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3 dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla legge 3 maggio 2004, n. 112. Ciò chiarito, sì fa presente che non si è mancato d'interessare, in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, la medesima RAI, la quale ha comunicato che la società SIGE (operante come *service* di ripresa, monitoraggio e trasmissione con la stazione ricevente della sede RAI di Palermo) collabora con la RAI dal 1991 tramite i suoi punti di trasmissione distribuiti sul territorio siciliano ed è stata sempre iscritta all'albo dei fornitori. Nel corso del 2005, in occasione della presentazione dell'aggiornamento dei dati societari per il mantenimento della suddetta iscrizione, sono emersi problemi che hanno portato alla momentanea sospensione del nominativo della società dall'albo. I problemi sono stati successivamente risolti con la presentazione di una nuova documentazione e da circa quattro mesi la medesima società risulta di nuovo regolarmente inserita nell'albo dei fornitori, per cui è stato possibile avviare le trattative per il rinnovo della convenzione tra la società RAI e la ripetuta SIGE. Nell'ambito di tali trattative vi sono state divergenze in merito al servizio da prestare e sui contenuti dell'intesa, che solo di recente sono state superate. Di conseguenza, il rinnovo degli accordi - stando a quanto riferito dalla stessa RAI - si trova attualmente in fase conclusiva. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il rappresentante del Governo per la tempestività con cui è stata fornita risposta all'interrogazione presentata da me solamente il 10 ottobre. una tempestività che mi auguro venga usata non solo nei confronti dell'interrogazione da me presentata, ma nei confronti di tutti senatori. Sarebbe buona abitudine, i rappresentanti del Governo rispondessero entro i termini previsti dal Regolamento. Detto questo, prendo atto della risposta non senza evidenziare però che alcuni elementi contenuti nell'interrogazione purtroppo non trovano

Prendo atto dalla risposta che il servizio è stato interrotto con la SIGE perché sono sorti problemi in ordine alla documentazione di cui i fornitori debbono disporre per mantenere l'iscrizione nell'albo dei fornitori. Il sottosegretario Vimercati sa bene che nell'interrogazione al riguardo ho indicato una causa precisa: sembrerebbe che il certificato di cui la ditta non disponeva fosse quello relativo ai requisiti antimafia o alla non sussistenza di reati a carico degli amministratori.

generica emersione di problemi, né capirei come tali problemi siano stati risolti in un tempo così breve, magari semplicemente modificando gli assetti societari della SIGE. Questo, comunque, non chiarirebbe le perplessità del sottoscritto. La seconda questione, che mi sono permesso di evidenziare, è legata al fatto che il rapporto tra la RAI e la SIGE è di per sé un problema.

il rapporto tra la RAI e la SIGE è di per sé un problema. Lo considera tale non solo l'USIGRAI, ma tutti i lavoratori RAI della Sicilia e lo considerano tale i siciliani, i quali hanno sempre individuato in questo rapporto, a partire dal 1991, uno dei punti di caduta della qualità del servizio radiotelevisivo pubblico in Sicilia. al periodo precedente al 1991, la RAI, intanto disponeva di una propria rete di ponti ad alta frequenza, che non si capisce perché doveva essere smantellata, e poi utilizzava per le riprese i cosiddetti operatori *free lance*,

che la stessa RAI utilizza. Dal 1991 tutto questo è scomparso. La RAI deve necessariamente rivolgere alla SIGE, che telefona agli stessi operatori *free lance* utilizzati dalla RAI in precedenza,

refluenze negative sulla qualità del servizio. Ma vi è di più: essendo la SIGE titolare di due reti televisive regionali ed avendo lo stesso rapporto anche con la concorrenza, Mediaset e La7, è del tutto evidente che i contenuti delle riprese venivano divulgati anche alla concorrenza e, talvolta, venivano utilizzati dalla stessa proprietà della SIGE per far concorrenza alla RAI. Quindi, io non credo che questa sia la soluzione migliore; ritengo che andrebbe, pertanto, rivisto complessivamente il modo con cui le immagini vengono trasmesse

mi dichiaro soddisfatto solo nell'ipotesi in cui il Governo si farà carico, per quanto di competenza, di chiedere alla RAI di riconsiderare la sua presenza in Sicilia e il suo rapporto con tale

La questione cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti è piuttosto complessa e delicata e concerne l'applicazione dell'articolo 8 della legge del 3 maggio 1999, n. Tale articolo ha posto a carico dello Stato il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed ha conseguentemente disposto il trasferimento nei ruoli statali di tutto il personale degli enti locali in servizio nelle scuole e negli istituti alla data di riferimento della legge, prevedendo l'inquadramento di questo personale nelle qualifiche funzionali

una procedura complessa che prevedeva tra l'altro - voglio sottolinearlo - la mancanza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Stato. Praticamente, i costi che lo Stato avrebbe dovuto affrontare per il personale entrato nei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai Comuni e alle Province da cui proveniva tale personale.

si fa riferimento ai criteri di inquadramento del personale interessato e, in particolare, al criterio del maturato economico: si collocano, cioè, gli interessati nella posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta *ad* *personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio. Ciò al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali (se superiore a quello dello Stato) nonché di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Per una completa conoscenza di questa complessa vicenda, è opportuno ricordare che le modalità di determinazione del trattamento economico per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali sono diverse. Infatti, per il personale statale la retribuzione è formata dal trattamento fondamentale - basato su classi di stipendio di importo progressivo, attribuite alla scadenza di periodi di servizio prestabiliti - nonché dal trattamento accessorio, disciplinato dalle norme contrattuali di settore; per il personale degli enti locali, invece, la retribuzione è formata dal trattamento economico fondamentale, cui corrisponde lo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità e dal trattamento accessorio, anch'esso disciplinato dalle norme contrattuali di settore. Quindi, diversamente dal personale del comparto scuola, per il personale degli enti locali - come avviene per la generalità degli altri dipendenti pubblici - l'anzianità di servizio è valutata a parte, con una specifica voce di stipendio che si aggiunge alle altre voci. Considerate tali differenze strutturali tra i trattamenti economici delle due categorie di personale, la disposizione dell'articolo 8 della legge n. 124 è stata applicata dall'amministrazione tenendo conto, ai fini dell'inquadramento nei ruoli statali del personale proveniente dagli enti locali, del trattamento economico complessivo in godimento che, come già detto, comprende anche l'anzianità di servizio - ed attribuendo agli interessati la corrispondente classe di stipendio prevista per il personale scolastico statale. Ho svolto questa complessa ricostruzione per indicare la complessità di queste equiparazioni e per dare conto anche di un altro aspetto: il diffuso contenzioso che si è determinato su questa vicenda e che si è concluso, in alcuni casi, in Corte di cassazione con la soccombenza dell'amministrazione centrale. Ma vi sono stati altri giudici che, in consapevole contrasto con la Cassazione, hanno espresso un diverso giudizio, condividendo le tesi dell'amministrazione, in in virtù della riconosciuta natura contrattuale dell'accordo del 20 luglio 2000 e della valenza, quale fonte normativa, di tale accordo. Su queste vicende è intervenuta poi la legge finanziaria 2006 che, all'articolo 1, comma 218, reca l'interpretazione autentica della norma Alla luce di questa norma interpretativa, risulterebbe quindi corretto il criterio di inquadramento adottato dall'amministrazione. Detto questo, convengo però con l'interrogante circa la situazione grave di disomogeneità nei trattamenti delle varie persone, che provengono da amministrazioni diverse, ma che oggi svolgono il medesimo ruolo. In questo momento, su questa vicenda complessa, pende il giudizio di illegittimità della Corte costituzionale sulla norma di interpretazione autentica; a questo giudizio che noi ci stiamo attenendo per le opportune valutazioni al riguardo. Io mi impegno, a nome del Ministero della pubblica istruzione e del Governo, a seguire con grande attenzione l'evolversi di questa situazione e ad assumere i provvedimenti conseguenti.

se il Parlamento intenderà affrontare, anche in sede di finanziaria, questa complessa situazione. Siamo anche noi molto preoccupati che si determinino e si consolidino condizioni di disparità di trattamento tra diversi dipendenti della pubblica amministrazione.

articolata e precisa ad un problema effettivamente complesso. Innanzi tutto mi dichiaro soddisfatto dell'impegno a seguire e a tener conto di eventuali proposte che il Parlamento volesse fare, anche nella prossima finanziaria. Dico subito, signora Vice Ministro, che io stesso presenterò, com'è stato già fatto alla Camera,

soddisfatto. Il tema, infatti, è complesso; certamente bisogna eliminare un *vulnus* (ecco il punto), quello che io ritengo un *blitz* - lo motiverò - della scorsa finanziaria, che ha tentato, in sede di interpretazione autentica, di passare sopra una legge, un accordo sindacale e pronunce giurisdizionali.

non si può fare se non si salvaguardano le condizioni dei lavoratori. Senza il contributo dei lavoratori, non si può riformare. Era giusta la legge: mettiamo nell'autonomia scolastica, sotto uno stesso punto decisionale, lavoratori provenienti da diverse amministrazioni, ma che lavoravano nelle stesse scuole. Il secondo tema i diritti dei lavoratori (diritti economici, ma anche di civiltà), il rilancio della scuola pubblica e l'uso improprio di una finanziaria per l'interpretazione autentica. Ovviamente, il mio emendamento tenderà semplicemente a ripristinare lo *status* Terza questione: il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. Non lo si può intendere - ecco la mia opinione di merito - solo come maturato economico, ma lo come anzianità di servizio. Infatti - lo ha detto con chiarezza la Vice Ministro - il maturato economico tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell'inquadramento nei ruoli statali, prescindendo dall'anzianità effettiva. Questo comporta un chiaro vantaggio per il personale all'inizio della carriera, il quale beneficia immediatamente dei miglioramenti retributivi e ha la prospettiva di beneficiarne a lungo per tutto lo svolgimento della prevista progressione economica, ma al tempo stesso provoca un appiattimento della posizione del personale con maggiore anzianità di servizio nell'ambito della medesima qualifica. Si crea effettivamente quella disparità di trattamento che lei stessa, signora Vice Ministro, richiamava. Da questo punto di vista,

che c'è un'«attribuzione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo goduto al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità». Insomma, è vero che si riconosce l'assegno *ad personam* - e ci mancava - ma si dà, di una questione chiara dal mio punto di vista della legge, nella quale i giudizi - come lei stessa ricordava - molto spesso hanno dato ragione ai lavoratori, un'interpretazione; peraltro, nel momento in cui il Parlamento votava, con una certa maggioranza,

né tanto meno si può accettare un trattamento differenziato all'interno del personale ATA, sfavorevole a tutti coloro che non hanno adito l'autorità giudiziaria o che non possono beneficiare di una sentenza passata in giudicato. É, quindi, necessario la norma *blitz* del 2005 venga superata: siamo fiduciosi che la nostra iniziativa, la sensibilità del nuovo Governo, che ringrazio ancora, e soprattutto l'iniziativa dei lavoratori che si stanno muovendo, porterà